Presidente, onorevoli colleghi, inizio il mio intervento esprimendo il cordoglio, mio personale e dell'intero Governo, per la tragedia avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 aprile nel Canale di Sicilia, nel corso della quale è affondato un barcone proveniente probabilmente dalla Libia e diretto verso l'isola di Lampedusa, con circa 200 persone a bordo. Fornisco i primi elementi acquisiti alla conoscenza del Governo, sulla base dei primi accertamenti. Le Forze armate maltesi hanno ricevuto, verso le ore 2,30 del 6 aprile, una richiesta di soccorso in mare per evento SAR, con cui s'intende la segnalazione di una imbarcazione in difficoltà e quindi la necessità di intervenire per fare *search and rescue*, ricerca e soccorso. La richiesta di intervento era partita da una persona che segnalava il possibile affondamento di un natante a causa delle avverse condizioni meteo marine. Le stesse autorità maltesi, che avrebbero dovuto intervenire, essendo l'area di competenza maltese, contattavano la centrale operativa della Capitaneria di porto di Roma richiedendo l'intervento delle autorità marittime italiane, dicendo che non avevano assetti navali disponibili. è già verificata in passato questa contesa senza senso tra Italia e Malta per l'intervento nelle aree di reciproca competenza. Abbiamo disposto l'invio delle nostre unità navali perché c'erano persone in difficoltà e ci è sembrato giusto, opportuno e utile soccorrerle prima di definire di chi fosse la competenza, perdendo tempo per scaricare su altri le responsabilità. Quindi, la Capitaneria di porto di Lampedusa metteva subito a disposizione due motovedette, un elicottero e un ricognitore aereo,

Nel corso dell'evento sono state salvate 51 persone, originarie del Centro-Africa, tra cui una donna e un neonato, che hanno detto di essere partite dalle coste della Libia. I superstiti hanno anche riferito che a bordo dell'imbarcazione erano presenti altre 150 persone, delle quali sono tutt'ora in corso le ricerche in mare, con l'ausilio anche di due navi mercantili; ma, ovviamente, più il tempo passa più le speranze di trovare altre persone in vita si affievoliscono. I superstiti sono stati ospitati presso l'ex base Loran di Lampedusa, alcuni di essi sono stati trasferiti presso le strutture ospedaliere dell'isola a causa delle precarie condizioni di salute. Anche in questo caso, pur non avendo alcun obbligo legale, le nostre forze

ma l'obbligo morale di salvare delle vite umane viene prima di qualunque altro dispositivo legale. Passiamo ai numeri. Dall'inizio dell'anno a oggi sono sbarcate 25.867 persone, in 390 sbarchi, 23.352 giunti nelle isole Pelagie (21.519 di questi di nazionalità tunisina); partiti dalla Libia sono invece 10 natanti, per un totale di 2.300 immigrati. È una distinzione importante, perché, come ha detto anche la commissaria europea, quelli che vengono dalla Tunisia sono migranti economici, e quindi senza i requisiti per essere considerati rifugiati o richiedenti asilo, mentre quelli che vengono dalla Libia sono

Abbiamo voluto investire in questo modello, perché riteniamo che l'assistenza per i rifugiati debba andare oltre la semplice accoglienza, e lì verranno svolte e sono già in corso attività di formazione, di insegnamento della lingua ed altre attività. Coinvolgendo anche le comunità locali, vogliamo che questo villaggio, che abbiamo nominato villaggio della solidarietà, possa essere un modello da portare in Europa. Abbiamo altresì investito sulla sicurezza attorno ai territori, firmando un patto per la sicurezza territoriale, a cui hanno aderito tutti i sindaci dell'area. Nonostante qualche tensione iniziale, che è avvenuta in tutti gli insediamenti

definizione di un patto territoriale per la sicurezza che coinvolge la Provincia di Catania e tutti i Comuni interessati. Questi 25.867 sbarchi hanno avuto la caratteristica di essere concentrati in pochissimi giorni; ciò ha causato una tensione straordinaria sulla piccola isola di Lampedusa, che ha determinato quelle condizioni di difficoltà di intervento che in altri casi, anche in presenza di dati numerici elevati, non si sono verificate negli anni passati. Qualcuno ha fatto riferimento ai circa 39.000 clandestini arrivati tra il 2008 e il 2009, prima che l'accordo con la Libia ponesse fine agli sbarchi dalla Libia, che purtroppo adesso sono ripresi per le condizioni di instabilità e di guerra in quel Paese.

quale era il motivo, e la loro destinazione: la stragrande maggioranza ha detto che è venuta in Italia per andare in altri Paesi, soprattutto in Francia. Questo ha creato - come avrete letto oggi sui giornali - qualche tensione con la Francia e con l'Europa. Per questo motivo, ci sarà un incontro bilaterale tra Francia e Italia il 26 aprile, la partecipazione del Presidente del Consiglio Berlusconi, del presidente Sarkozy, dei Ministri dell'interno e dei Ministri dell'economia. Credo che la cosa più sbagliata sia quella di farci la guerra tra di noi: se l'Europa è davvero un soggetto che vuole giocare un ruolo politico e di integrazione, prima di tutto tra i Paesi, dobbiamo trovare una soluzione che sia una soluzione europea. Lo dirò e lo ribadirò nel corso del mio intervento: è il ruolo che finora è mancato, e non per incapacità o cattiva volontà di chi governa la Commissione; anzi, il commissario europeo Cecilia Malmström è sempre stata in contatto con me sin dall'inizio, esprimendo la totale disponibilità a far ciò che è di sua competenza, che purtroppo però è molto poco, se non la disponibilità a risarcire l'Italia con un fondo di 25 milioni di euro, da suddividere peraltro tra i 27 Paesi europei, o un rafforzamento dell'attività di coordinamento dell'Agenzia Tutto il peso della gestione di questa emergenza, sia nel Mediterraneo sia a Lampedusa, anche successivamente, è stato esclusivamente sulle nostre spalle. È una vicenda che ci deve insegnare, e deve insegnare all'Europa, che, di fronte a questo sommovimento nei Paesi del Maghreb, non è sufficiente che l'azione di contrasto all'immigrazione clandestina sia lasciata agli Stati rivieraschi e solo sul fronte del controllo dell'immigrazione clandestina. È una vicenda più complessa, ne vanno rimosse le cause, e solo un ruolo più attivo dell'Europa nella prevenzione di questi fenomeni,

e i mezzi necessari per far fronte a questa concentrazione di sbarchi in pochissimi giorni, che hanno determinato una condizione molto dura anche e soprattutto per i cittadini di Lampedusa, che ringrazio per la pazienza e l'aiuto che hanno dato. Il Consiglio dei ministri, come sapete, ha incaricato l'onorevole Sonia Viale, insieme ad altri, di definire un piano di interventi compensativi

spostare queste persone in strutture di emergenza, che si sono rese necessarie proprio per l'intensità e la concentrazione degli sbarchi in pochissimi giorni. Strutture di emergenza, centri di prima accoglienza che abbiamo organizzato in alcune località - e poi dirò dove - proprio per tamponare la situazione e dare un ricovero adeguato a queste persone, cosa che è avvenuta, e per procedere all'identificazione

Sono stati allestiti a Trapani nell'ex pista aeroportuale dell'Aeronautica militare, a Caltanissetta nei pressi del CARA di Pian del Lago, a Mineo nel già citato Residence degli aranci, a Manduria in Puglia (un centro di prima accoglienza), a Potenza in località località Piani di Palazzo San Gervasio, a Santa Maria Capua Vetere presso la caserma «Fornaci e Parisi», a Civitavecchia presso la caserma «De Carolis», in Molise, a Campochiaro presso il centro funzionale del servizio regionale di protezione civile, a Cagliari presso la caserma di via Elmas e a Ventimiglia (come centro di prima accoglienza). In Toscana è stato definito, d'intesa con il Presidente della Regione, un dispositivo diverso. La Regione ha individuato, in cooperazione con il Ministero dell'interno, 11 siti, per una capienza complessiva di circa cinquecento persone. È un modello diverso dagli altri che abbiamo allestito, un modello interessante, che ho riconosciuto e che può essere utilizzato terminata la fase acuta dell'emergenza che ci ha costretto a realizzare questi siti temporanei per far fronte ad una concentrazione di sbarchi in pochissimi giorni. Abbiamo assunto subito una serie di iniziative su tre fronti: il fronte interno, con le Regioni e gli enti locali, il fronte europeo e, naturalmente, i Paesi di provenienza degli immigrati. Sul fronte interno, abbiamo coinvolto le Regioni e gli enti locali in una serie di incontri per definire le misure necessarie per

un intervento per distribuire su tutto il territorio nazionale, secondo criteri legati alla popolazione, in tutte le Regioni, escluso l'Abruzzo, un numero fino a 50.000 tra profughi e rifugiati. Fino ad oggi sono 2.300

riguardato un'imbarcazione partita dalle coste libiche, da quelle stesse località da cui fino al maggio del 2009 i trafficanti di esseri umani facevano partire i barconi. Dal maggio 2009, a seguito

Accanto a questi ci sono coloro che sono arrivati dalla Tunisia. Nell'accordo con le Regioni del 30 marzo si parlava anche del problema dei minori stranieri non accompagnati.

che non saranno rimpatriati, in quanto minori, neanche se vengono dalla Tunisia, sono stati affidati alle case famiglia attraverso i Comuni. sono partiti tra ieri e oggi. Non c'è un ritardo: è che la procedura prevede l'individuazione delle strutture in cui metterli, il coinvolgimento dei Comuni e il controllo, come è giusto che sia, dell'autorità giudiziaria, senza il nulla osta della quale non possono essere trasferiti da Lampedusa. Sono stati accelerati i tempi anche da parte dell'autorità giudiziaria, e gli ultimi minori sono stati trasferiti.

e che oggi sui giornali appare un po' come una novità, ma che tale non è. Si tratta cioè dell'attuazione, anche per quanto riguarda gli immigrati, quindi non i rifugiati, di un criterio di equa e sostenibile attribuzione,

applicato forse in modo più efficace rispetto alla fase che abbiamo gestito finora, che però, lo ripeto, era di emergenza acuta, perché in pochi giorni abbiamo dovuto trasferire 25.000 persone.

anche il tema dell'emergenza umanitaria che noi abbiamo da subito individuato, emanando anche, come sapete, una ordinanza per l'emergenza umanitaria e incaricando il prefetto di Palermo Caruso della gestione di una situazione molto difficile e complicata. Voglio pubblicamente pubblicamente ringraziare il prefetto Caruso per lo straordinario impegno che ha profuso e, assieme a lui, le forze dell'ordine (la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di finanza e i Vigili del fuoco) che hanno dimostrato un'eccezionale professionalità nella gestione di questo

non so quando potranno essere conclusi. Peraltro, c'è il problema politico che la maggioranza degli Stati europei è contraria e ha già dichiarato la sua contrarietà, alla attivazione della direttiva. Perché? Perché l'attivazione della direttiva significa l'applicazione di quel principio che il Governo italiano sostiene da tempo in materia di profughi e non solo, e cioè della condivisione degli oneri della redistribuzione di queste persone sull'intero territorio europeo in base a criteri da definire, il cosiddetto *burden sharing*, principio al quale si oppongono molti Paesi europei.

il sistema europeo comune di asilo da realizzare entro il 2012: siamo lontanissimi da questo, perché c'è il veto di alcuni Paesi europei (Inghilterra in primo luogo); Paesi che non mancano di ricordare all'Italia i doveri di attuazione e applicazione dei principi generali, dei criteri di assistenza, di umanità e così via, ma che poi, quando si tratta di condividerne gli oneri,

La difficoltà deriva dall'ostilità che al principio della condivisione degli oneri derivanti dalla immigrazione nei Paesi di confine viene opposta dai Paesi che di confine non sono. È un brutto esempio di ciò che l'Europa dovrebbe essere e non è. Penso che la scelta di lasciare

un residuo di sovranità che consente agli Stati di decidere le politiche sull'immigrazione all'interno del proprio confine. Tuttavia, questo contraddice il principio della libera circolazione nei Paesi, almeno di area Schengen, e quindi è opportuno che a partire da questo fenomeno detto e ribadisco, di immigrazione clandestina, bensì di movimenti di massa che ancora non si sono manifestati nella loro complessità

gestire il rapporto con i Paesi extraeuropei, in particolare con quelli del Nord Africa, al fine di prevenire i fenomeni. Abbiamo stipulato un accordo un accordo con la Tunisia per il contrasto all'immigrazione clandestina, ma è ovvio che occorre intervenire sulle cause attraverso politiche di cooperazione internazionale che impediscano ad un'intera generazione - perché di questo parliamo - di giovani tunisini di abbandonare il proprio Paese per l'impossibilità di crearsi una vita come si deve.

da parte tunisina è sempre stato interpretato in modo molto restrittivo, prevede la possibilità di rimpatriare non più di 3-4 cittadini al giorno, anche se i numeri sono molto più elevati.

20.000 cittadini tunisini, l'anno scorso ne erano arrivati 25 (in tre mesi). Quindi, anche il rimpatrio di 3-4 cittadini al giorno si poteva gestire bene. Quest'anno c'è qualche problema in più. È per questo che, oltre all'accordo del 1998 e all'accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità del dicembre 2003, che ho rinnovato e aggiornato nel gennaio 2009, abbiamo

con l'intervento del Ministero degli esteri in materia di cooperazione di sicurezza. L'accordo che ho sottoscritto prevede alcune iniziative, in particolare mirate alla prevenzione dei flussi e al rimpatrio dei cittadini tunisini che arriveranno dalla sua firma in poi. L'oggetto della cooperazione è quello di rafforzare la collaborazione tra le forze di sicurezza italiane e tunisine al fine di prevenire gli sbarchi di clandestini verso le coste italiane (è quanto si legge nel testo dell'accordo), intensificare la lotta all'immigrazione irregolare e alla tratta di esseri umani, assicurare la protezione e la salvaguardia delle vite in mare. Prevede procedure di rimpatri semplificate: l'Italia e la Tunisia concordano sul rimpatrio di tutti i cittadini tunisini che arriveranno in Italia dopo che l'autorità consolare tunisina ne avrà accertato la cittadinanza, sulla base di procedure semplificate e quindi rapide. Ancora più importante è la cooperazione operativa per prevenire questi fenomeni: aumentare i controlli, rafforzare la sorveglianza, l'intervento e il soccorso sia in mare sia in mare che sulla terra (dove oggi questi controlli sono praticamente svaniti) attraverso lo scambio in tempo reale di ogni informazione utile, la fornitura di strumenti necessari,

Il personale delle forze di sicurezza dell'Italia e della Tunisia parteciperà alle attività di formazione in materia di sorveglianza marittima ed aerea, di contrasto all'immigrazione irregolare e

e allo scambio di personale di coordinamento (ufficiali di collegamento), fino a questo momento assente, per rafforzare il sistema di cooperazione. Questo accordo è molto importante perché definisce le procedure, le modalità e gli strumenti per contrastare efficacemente l'immigrazione clandestina. Naturalmente, adesso

Abbiamo quindi gestito la questione interna nel rapporto con le Regioni e gli enti locali. In merito alla questione del rapporto con i Paesi rivieraschi, funzionano bene gli accordi con l'Egitto, l'Algeria e il Marocco. Con la Tunisia, questo nuovo accordo apre prospettive molto interessanti, ma il fronte europeo è quello che abbiamo aperto, e che merita un'attenzione ed un'azione molto intensa. Su questo, contiamo

I nuovi assetti dell'area del Maghreb e di quella del Medio Oriente sono in corso di definizione. Può succedere che tutto si stabilizzi, ma può succedere anche il contrario. Credo che la visione miope finora proposta

con una visione più ampia e lungimirante, politiche di intervento proattivo nei confronti dei Paesi in questione. Sul fronte della cooperazione internazionale - come ho già detto - è questo il sistema per prevenire i flussi migratori irregolari; di questo si è fatto carico il Presidente del Consiglio, che al Consiglio europeo ha sottoposto la questione; di questo ci faremo carico nell'incontro tra la delegazione italiana e quella francese, fissato ai massimi livelli il 26 aprile presidenti Berlusconi e Sarkozy e numerosi Ministri. Questa è la dimensione europea che finora è mancata e che noi abbiamo chiesto, oltre a quella dell'accoglienza o del principio del *burden sharing*: una politica attiva che superi

diversificato di cui i trafficanti di esseri umani approfittano, mandando di qui piuttosto che di là cittadini di quelle nazionalità, sapendo che sulla base degli accordi bilaterali possono essere rimpatriati o meno. Si tratta una situazione nata per talune ragioni, ma che oggi non è più attuale e deve essere modificata. Occorre che l'Europa assuma un ruolo come Unione europea per definire accordi bilaterali: da una parte l'Europa, dall'altra i vari Paesi extraeuropei, È una sollecitazione forte che abbiamo fatto; qualcosa si sta muovendo. Il presidente Barroso è in contatto con il presidente Berlusconi su questo punto specifico; mi auguro davvero che, anche che, anche grazie all'esperienza che l'Italia ha maturato in tutti questi anni, e che mettiamo a disposizione dell'Unione europea, si possa aumentare la velocità di reazione dell'Unione europea, che finora è stata assolutamente troppo troppo lenta, lasciando all'Italia, e solo all'Italia, il carico esclusivo della gestione di un'emergenza umanitaria così complessa, così difficile e così

intraprendere un'azione comune. Da ultimo, l'accordo con la Tunisia prevede che da oggi in avanti coloro che arrivano vengano rimpatriati. Oggi il Presidente del Consiglio firmerà il

i requisiti di sicurezza. Saranno esclusi coloro che sono stati riconosciuti appartenere a categorie socialmente pericolose (quelle di cui

ancora efficace; coloro che risultino denunciati o essere stati detenuti nelle carceri tunisine per una serie di reati. Chi rientra in queste categorie non avrà, naturalmente, il premesso di soggiorno per fini umanitari e sarà messo nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) per poter essere poi rimpatriato in Tunisia. Tale permesso di soggiorno consente all'interessato la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea, come previsto dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Come ho detto, la stragrande maggioranza degli intervistati ha detto di voler andare nei Paesi europei,

tra Italia e Francia, e non solo per gestire questo fenomeno. Finora purtroppo la reazione del Governo e del sistema francese è stata di ostilità: non credo che questo sia un buon atteggiamento, anche perché la libera circolazione è garantita nell'area Schengen da regole che devono essere applicate, e di questo discuteremo il 26 aprile con il presidente Sarkozy.

sono un atteggiamento e una prospettiva diversi: rimane l'emergenza umanitaria, ma possiamo dire che si apre una fase nuova, che potrà portare a risultati di contrasto all'immigrazione clandestina, come tutti ci auguriamo che avvenga con l'attuazione dell'accordo con la Tunisia, e a una maggiore responsabilizzazione dei Paesi europei, che finora non c'è stata.

desidero innanzitutto associarmi alle parole di cordoglio da lei pronunciate all'inizio di questa nostra seduta per le vittime e per i dispersi dell'ultima di una lunga, triste serie

in cambio della circostanza che rapidamente il Governo tunisino - che attraversa una fase di crisi dovuta alla vicenda della fuga del suo Presidente Ben

si tratta cioè di profughi, ossia gente che è scappata da quel Paese e che oggi - perché non è operativo il Trattato con la Libia - ha la possibilità di vedere riconosciuto, quando riesce ad arrivare in Italia o in Europa, il proprio *status* di rifugiato. Fino a ieri, l'accordo con il leader Gheddafi e il trattato che questa maggioranza e questo Governo hanno approvato in questo Parlamento hanno fatto di tutta un'erba un fascio, mischiando i migranti clandestini che passavano dalla Libia con gli eritrei e quanti altri si sono trovati costretti a fuggire dalla propria terra. Purtroppo, oggi le lacrime da coccodrillo non servono a niente, perché quelle vittime sono purtroppo la testimonianza del fallimento di una politica estera del nostro Governo che ha puntato tutte le proprie carte sul rapporto con Gheddafi e ha perso, ha sbagliato. Se oggi il Ministro degli affari esteri ha dovuto dichiarare che bisogna superare la fase relativa a Gheddafi in Libia ed ha riconosciuto - come peraltro tante forze politiche in questo Parlamento gli hanno chiesto - le forze di opposizione al dittatore libico, è perché ha dovuto prendere atto che tutto quello che fino ad oggi questo Governo ha fatto in materia di politica estera è tragicamente sbagliato. Signor Ministro, abbiamo ascoltato le sue parole

nei confronti della nostra Marina militare, che da sempre opera nel Mediterraneo e salva vite umane, l'apprezzamento nei confronti delle forze dell'ordine e del volontariato. Ma senza di esse, senza il volontariato o la Marina militare, il nostro Paese avrebbe fatto una figura ancor peggiore di quella che le immagini di Lampedusa hanno trasmesso in tutto il mondo. E di questo, signor Ministro, non credo che né lei né noi possiamo andare La verità è che voi avete commesso un errore: quello di pensare di affrontare una situazione eccezionale in maniera ordinaria o, peggio ancora,

che ha fatto del reato di immigrazione clandestina la madre tutte le battaglie e la panacea di tutti i mali della immigrazione irregolare. Ebbene, oggi possiamo dire, signor Ministro - mi scusi se la disturbo - che l'adozione tardiva del decreto col quale si riconosce si riconosce la protezione umanitaria ad oltre 25.000 migranti,

Si tratta di una sanatoria resasi necessaria per evitare che il tribunale di Agrigento aprisse 25.000 procedimenti penali per immigrazione clandestina. Si tratta di una sanatoria per evitare che questi migranti, che in parte hanno la necessità di transitare in altri Paesi dell'Unione europea, vedessero chiusa la frontiera francese a Ventimiglia, così come è stato in questi giorni. Però, siamo convinti che non si tratti di una sanatoria - mi dispiace doverlo dire ai colleghi della Lega - ma - ma di un provvedimento che tardivamente è stato adottato dal Governo per ragioni politiche e non oggettive. Tardivamente è stato utilizzato dal Governo, perché questo provvedimento, signor Ministro, le consente di attivare la direttiva 2001/55/CE, che stimola il Consiglio europeo a riconoscere che l'emergenza umanitaria debba essere condivisa da tutti gli Stati dell'Unione perché quella direttiva, non quella che non volete e non sapete recepire, cioè l'ultima sui rimpatri, già abilita gli Stati membri a farsi carico della propria responsabilità ai fini della protezione umanitaria. Questo decreto serve sostanzialmente anche a questo, se lo volete fare e se avete l'autorevolezza e la credibilità internazionale per poterlo fare; rinvio agli articoli 4 e seguenti della direttiva 2001/55/CE. Di questo dobbiamo parlare, del ritardo con cui questi problemi sono stati affrontati. Voglio aggiungere anche che la infelice dichiarazione del suo ministro Bossi, «fora de ball», ha fatto più danni di tanta politica estera degli ultimi anni. Se c'è stato un irrigidimento anche del Governo tunisino è dovuto al trattamento che noi abbiamo riservato con la nostra insipienza ai tunisini a Lampedusa e alla circostanza che questo trattamento, al di fuori di ogni minima logica di garanzie e di rispetto dei diritti umani - non parliamo poi della protezione per donne e bambini ha inasprito anche quelle frange più estremistiche che in Tunisia ci sono e sono il vero pericolo per la stabilità politica di quella democrazia che si sta costruendo.

perché ancora fate confusione tra clandestini e profughi e perché il sistema eccezionale è in realtà, dal punto di vista quantitativo, di gran lunga inferiore ad altre ondate migratorie emergenziali che questo Paese ha vissuto, ad esempio dai Balcani

sull'improvvisazione della distribuzione territoriale dei migranti con le tendopoli, che non fanno onore ad un Paese civile, testimoniano che la Sicilia ha pagato e continua a pagare il prezzo più alto, che il Mezzogiorno ha pagato e continua a pagare il prezzo più alto e che fino alle prossime elezioni amministrative lei non può spiegare al suo partito che al Nord si devono fare dei centri di accoglienza. Quando ci fornirà i dati su come, dove e quando questi centri verranno aperti anche in Lombardia, Veneto e Piemonte, la sua politica e le sue dichiarazioni di grande solidarietà saranno credibili. Fino a quel momento valgono le parole del suo sottosegretario, l'onorevole Mantovano,

che il cambio di atteggiamento di questi giorni da parte vostra testimonia che avete sbagliato e che volete cambiare rotta.

Gli spettacoli cui abbiamo assistito in televisione non fanno onore a un Paese civile come il nostro e a un Governo che deve abbandonare la linea del populismo, perché non serve a niente ed è fallimentare nel contrasto all'immigrazione clandestina.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ci chiediamo se ci sono dei colpevoli, degli assassini delle centinaia di persone che sono tragicamente annegate nel Canale di Sicilia, a cui lei, offerto la solidarietà profonda del nostro Senato. Una risposta è necessaria, e siamo in grado di darla. In troppi maledicono il mare o la scarsa umanità di qualche Governo, ma gli assassini hanno una precisa identità: sono le organizzazioni criminali che trafficano gli esseri umani. Stiamo facendo abbastanza per contrastarle? No. Stiamo predisponendo misure per modificare questa situazione? Assolutamente no. Il ministro Maroni ci ha dato una comunicazione corretta sui fatti, ma del tutto reticente sulle motivazioni dei fatti e sugli errori capitali commessi dal Governo.

Cinque errori capitali che sono conseguenza delle pretese demagogiche, presuntuose e pretestuose della Lega. Primo. Il Governo non ha predisposto per tempo - nonostante fosse previsto ed annunciato da lei stesso, un mese fa, l'arrivo di migliaia di migranti - un piano nazionale per il loro smistamento, determinando la drammatica crisi di Lampedusa. Secondo. Esplosa la crisi, il Governo ha ripartito i flussi in modo smaccatamente irresponsabile - tutti subito in Sicilia e nelle Regioni del Sud - provocando così le dimissioni del sottosegretario Mantovano, cui lei non ha dedicato neppure una parola. Terzo. Ha rifiutato di prendere in esame l'applicazione dell'articolo 20 del Testo unico sull'immigrazione, che permette la protezione umanitaria con permessi temporanei. Anche questa è una scelta strettamente ideologica. Quarto. Questo ritardo ha creato il caos al confine italo-francese ed ha allontanato la possibilità, signor Presidente, dell'assunzione di maggiori responsabilità da parte dell'Unione europea, visto che tra queste persone vi sono richiedenti asilo, cui l'Italia deve prestare protezione, lo sottolineo, ma anche molte persone che mirano a raggiungere altri Paesi europei. Apro una parentesi, signor Ministro, su quello che lei ha definito il *partner* *sharing*, cioè la ripartizione di responsabilità: ma con che credibilità vi presentate in Europa, voi che vi caratterizzate per lo *slogan*: «Fuori dalle balle»? Con che credibilità vi presentate a dialogare con gli altri Ministri europei? Ma lo sa, signor Ministro, che la Germania ha assunto centinaia di migliaia di rifugiati? Lei è andato in Tunisia, e sa benissimo che i tunisini hanno il problema delle centinaia di migliaia di rifugiati che attraversano l'ormai incontrollato confine con la Libia. Voi parlate in termini demagogici, privi di concretezza e pretendete che l'Europa, che insultate quotidianamente, assuma le responsabilità che spettano all'Italia nella cornice europea. Ora, signor Presidente, è evidente, ed è il quinto punto fondamentale su cui centrerò la parte finale del mio intervento, che il Governo continua a sottovalutare l'incidenza strategica del traffico di persone sul piano umanitario e per la sicurezza nazionale. precise proposte che un rapporto del COPASIR, approvato all'unanimità nel 2009, ha formulato in Parlamento. Oggi, Presidente, la crisi totale della cornice di sicurezza e di controllo tra Libia e Tunisia è il problema. Ci si illude di limitare fenomeni giganteschi dentro i 20 chilometri quadrati dell'isola di Lampedusa o altrove? Intendiamo mettere alla prova, signor Ministro, alcuni suoi annunci: oggi stesso presenteremo una mozione al Senato perché l'Italia assuma una *leadership* europea e internazionale sul piano umanitario, della prevenzione e del contrasto al traffico di esseri umani. Siamo potenzialmente la porta d'accesso porta d'accesso per milioni di disperati e di persone desiderose di migliorare le proprie condizioni di vita. Queste persone, Presidente, non arrivano attraverso i ben noti percorsi del Golfo di Guinea o dal Corno d'Africa, acquistando un biglietto del treno o dell'autobus. Questa spinta umana, che può diventare travolgente, è attivata da organizzazioni e reti criminali che stanno realizzando grandi guadagni, e dunque si stanno ulteriormente rafforzando. Il nostro Governo ha le mani legate: sì,

alla perdita di autorevolezza internazionale e all'incapacità gestionale delle crisi umanitarie, noi chiediamo la formazione di un altro Governo, non inchiodato alla propaganda, ma capace di affrontare i grandi problemi del nostro

per essersi ancora una volta dimostrato in grado di affrontare difficoltà di portata storica non facilmente superabili. La ringrazio per tutto ciò che ha fatto e, in ultimo, per l'accordo raggiunto con la Tunisia, che auspico fortemente possa ricondurre la situazione verso la normalità. Ringrazio anche il presidente Berlusconi per l'impegno e la determinazione verso i cittadini di Lampedusa. Non ho mai voluto strumentalizzare in tutti questi anni l'invasione degli immigrati per ottenere cose che spettano di diritto alla mia isola. da molto tempo Lampedusa vive direttamente la costante emergenza degli sbarchi di immigrati clandestini e le tragedie umane connesse a questo fenomeno, ma questa volta, credetemi, la situazione ha assunto dimensioni ben più drammatiche nella realtà di quelle che le immagini televisive hanno potuto mostrare. Gli abitanti di Lampedusa hanno affrontato questa emergenza straordinaria con grande coraggio, dimostrando un'umanità e una disponibilità che merita riconoscenza, ma soprattutto merita da parte del Governo la ferma determinazione a cercare soluzioni durature per quest'isola, che resta territorio di confine tra due mondi, ma che appartiene al nostro Paese e all'Europa. Se per ipocrisia e strumentalizzazione politica contro questo Governo si sottovaluta la portata del problema dell'immigrazione illegale, di fatto si incoraggiano gli esodi di massa, cari colleghi di sinistra, e si ingenerano aspettative, alimentando la spirale delle sofferenze, che ricordiamo indistintamente, su tutti e e su tutto il nostro Paese. Siamo tutti consapevoli e fiduciosi che questo Governo, questo Ministro dell'interno, continuerà costantemente a trovare le risposte più giuste nell'interesse collettivo, soprattutto quelle coerenti con la determinazione a far rispettare la legalità e a difendere i nostri diritti. E lo farà, anche se sappiamo che chi lotta per i propri princìpi si espone alle critiche di quelli che offrono soluzioni facili e demagogiche,

vorrei commentare alcune cose di questi giorni in maniera più tecnica per addetti ai lavori, nella speranza che qualcuno impari. Il flusso di rifugiati dai Paesi del Maghreb sarà sempre più massiccio in futuro, non solamente dalla Tunisia, ma da tutti i Paesi africani che abbiano situazioni di grave crisi economica o di guerra (al momento 9, ma per quest'anno Forse l'Italia e il Governo italiano non se ne sono accorti. Parlare di 60 ore per ripulire Lampedusa, oppure fare proclami che fanno piangere, e non più sorridere,

crisi sì o crisi no; Libia, Egitto o altri Paesi. Il problema vero sta nel non aver capito, da anni, che è inutile continuare a parlare di emergenze. I Governi italiani che si alternano da tempo parlano sempre e solo di emergenze, mai di prevenzione e di investimenti nella prevenzione. Chi dovrebbe lavorare, unitamente a colleghi che operano a livello internazionale, incessantemente, fa viaggi e pensa ai fasti del passato, speso male, con i soldi degli italiani. Con i soldi che invece spenderemo ora, avremmo potuto lastricare d'oro i centri d'accoglienza e farli divenire centri d'eccellenza di fronte all'Europa e al mondo, con facilitatori e mediatori linguistici, con *training* per posti di lavoro e corsi di lingua italiana per chi desidera rimanere a lavorare nel nostro Paese, con diritti e doveri, come in altri Paesi. Le comunità locali avrebbero potuto diventare una risorsa, avremmo potuto creare posti di lavoro proprio lì dove questi centri vengono creati. Anche un centro di espulsione necessita di personale. Nessuno in Europa ha risolto i problemi dell'immigrazione. Nessuno ha risolto un problema di queste dimensioni, che sarà sempre più grande. Il decreto permessi temporanei non risolverà il problema dei flussi migratori, il problema dei flussi migratori, che interessa intere regioni del mondo, e non dell'Italia, con milioni di persone. L'immigrazione può determinare il cambiamento di un tessuto sociale di un intero Paese. Non illudiamoci di risolvere tutto con permessi temporanei, sanatorie, emergenze. È ora di affrontare il tema in termini strategici. Siamo in ritardo di 20 anni. Non ci illudiamo di risolvere questo problema dall'oggi al domani, come stiamo facendo.

Bisogna cominciare ora a pensare al medio e al lungo termine per essere artefici del futuro della società italiana. Bisogna cominciare a pensare ad un Governo che sia più attento non solo a quello che succede all'interno del nostro Paese. Non siamo soli.

La nostra politica estera è assente da anni, e i fatti di questi ultimi giorni non fanno che dimostrare che è cosi. Le corse all'estero per cercare soluzioni lo dimostrano. Fare tutto di corsa non va bene: vuol dire che non si è capito nulla. è un Governo distratto, signor Ministro. Il Presidente francese non verrà di corsa il 26 aprile. Non mi sembra che corra per il 26 aprile. In 20 giorni cambia il mondo, quando un Paese è in guerra o c'è una crisi. La prova del fallimento italiano in politica estera è la fine annunciata del nostro prestigio internazionale, per non parlare dei colleghi parlamentari tunisini che hanno dato lezioni, infine evitando la vergogna per la nostra presa di posizione su Bengasi. Il problema è nostro. Dovevamo avere una politica estera lungimirante e previdente. Dovevamo provarci, e noi non ci abbiamo neanche provato.

la corsa dei nostri Ministri, la non corsa di Sarkozy, la vittoria del Governo tunisino ai danni dell'Italia, conclamata dai *media,* lo spreco enorme di risorse,

persone in attesa di *status* di rifugiato da mezza Italia, confinandole nel mezzo di una pianura deserta, sia le commissioni territoriali, magari creandone una nuova, quindi azzerando tutti processi di richiesta di *status* di rifugiato.

Una circolare che non è stata neanche resa nota agli interessati, cioè ai parlamentari e ai consiglieri regionali, che potrebbero fare visite ispettive, perché sicuramente in questi luoghi, organizzati in poco tempo, le situazioni di convivenza e le condizioni igienico-sanitarie sono di grave crisi.

recepimento della direttiva rimpatri. Non si capisce infatti come mai un ulteriore strumento di norma a livello europeo sia stato respinto in un momento in cui già si sapeva che si sarebbero verificate presenze sempre maggiori. Ci è stato poi evidenziato un terzo fronte, che sarebbe quello dei Paesi di provenienza, con i quali si sta cercando di concludere dei trattati. Se fossero veri i contenuti apparsi poco fa sul sito del «Corriere della Sera» relativamente a quello raggiunto con la Tunisia, si parla soltanto di *computer*, jeep e altre strumentazioni di tipo meramente paramilitare, per evitare che queste persone partano. Occorre investire in promozione della democrazia, in promozione e sviluppo economico, quindi recuperando tutti i tagli fatti alla cooperazione internazionale, perché non si può continuare a gestire il tutto come se fosse esclusivamente un problema di ordine pubblico. Sono stati dati molti numeri, e l'ultimo è quello di 2.300 persone provenienti dalla Libia che potrebbero essere pronte per ricevere lo *status* di rifugiato. Ecco, occorre stare molto attenti, ma, ripeto, più che valorizzare Mineo, occorre valorizzare il modello Toscana, perché la distribuzione sul territorio di pochi numeri per varie Province è sicuramente il modello che può cercare di farci recuperare un minimo di credibilità di fronte agli europei. Un'ultima questione: il Ministero degli interni francese da poche ore ha pubblicato sul sul sito cinque punti per i quali saranno pronti ad accogliere eventuali accordi con l'Italia. Da qui al 26, cioè tra tre settimane, spero che l'Italia almeno faccia conoscere in maniera dettagliata ciò che sta portando avanti a livello bilaterale con il resto dei Paesi coinvolti in questa crisi.

perché, con molto garbo devo dire, il funzionario della Questura mi spiegò in quel momento che c'erano problemi di disordine: ritengo che noi parlamentari dobbiamo eventualmente andare a visionare queste situazioni non certo per creare ulteriore disordine, ma per essere semplicemente di

a difendere le ragioni dell'Italia. Lo trovo profondamente ingiusto nei suoi riguardi perché anch'io personalmente la apprezzo molto, e non mi sembra che un Ministro della Lega debba assumersi da solo, fino in fondo, le responsabilità di quanto è accaduto. Trovo che le manchi accanto qualche altro rappresentante del Governo. Lei oggi ha ricordato gli Esteri e la Difesa, ha detto di avere organizzato un intergruppo (non so, sarà penso che le sia molto mancato un supporto per quello che potesse riguardare le politiche comunitarie: manca un Ministro per le politiche europee da troppo tempo. Manca un Ministro, quindi, che abbia realmente rapporti con l'Europa per indurre quell'Europa, che lei giustamente ha ricordato tante volte, a fare innanzitutto il suo mestiere, a non essere più ipocrita ed egoista come quell'Europa che pretende dagli Stati membri che applichino le direttive europee mentre poi essa stessa si tiene ben distante dall'applicazione delle medesime direttive, Trattato di Schengen ha necessità ancora di essere interpretato, e non invece semplicemente applicato. no? - la Protezione civile, le è mancato il Bertolaso di turno, qualcuno che le venisse incontro in questo momento; le è mancata una vera politica regionale,

come altro definirli, se sfollati, persone che hanno diritto al rifugio o all'asilo, quel che sia. Diciamo: gente, povera gente, che sta morendo nel Canale di Sicilia, e per la quale tutti noi, solidalmente, piangiamo, ma rispetto alla quale non siamo stati capaci di fare assolutamente assolutamente nulla). Le Regioni, signor Ministro, dovrebbero assumere fin d'ora una sorta di regolamento, di patto

anche cittadini europei. Non abbiamo mai lo spirito comunitario. Parliamo e blateriamo di sussidiarietà verticale, ma quando si tratta di applicarla all'interno del nostro Stato non sappiamo neanche di che cosa realmente stiamo parlando.

e cosa devono fare gli Stati. Se ho ben compreso da quel che lei ha riferito, signor Ministro, mi sembra molto strano che oggi si debba chiedere all'Europa cosa si debba fare in base a quella direttiva e se e come gli Stati la possono applicare. Gli Stati dovevano recepirla entro la fine del 2002. L'Italia l'ha recepita all'inizio del 2003 con una legge nella quale ha scritto delle cose; ma anche gli altri Stati

sarebbe trattato di un sistema comunitario di sussidiarietà in virtù del quale i singoli Stati si sarebbero dovuti assumere le loro responsabilità.

un'emergenza che va spalmata su tutta l'Italia. Non intendo fare polemica neanche sulle frasi ad effetto, perché - le conosciamo tutti - può averle dette Bossi, come le ha dette Vendola, il quale, da presidente della Regione Puglia, invece di fare qualcosa qualcosa per la sua regione, ha pensato bene di fare un comizio splendido a Manduria, che non è servito assolutamente a nessuno, ma semplicemente a fomentare gli animi e a creare quegli elementi di conflitto

a creare conflitti, bensì a far partecipare questa gente alla vita democratica della città. Questo, per far comprendere le regole, per informarli sui diritti, ma anche per pretendere i doveri di civile convivenza all'interno della mia città. C'è stata - signor Ministro, mi consenta di ricordare anche questo - una mancanza rispetto alla cooperazione allo sviluppo. Da ex deputato me ne è buona testimone - qual è il mestiere esatto di tante organizzazioni non governative che prendono, per dirla fuori dai denti, un sacco di

Italia è aumentata e non è diminuita, allora significa che qualcosa non ha funzionato: significa che qualcuno ha preso del denaro, ma non ha investito

Ministro, le chiedo che si faccia non solo un'informativa - lei l'ha fatta in maniera misurata, e personalmente le sono

riesce mai a guardare con molta attenzione.

alle famiglie delle povere vittime di una tragedia immane che, negli ultimi tre mesi - secondo una ricostruzione pubblicata su tutti i giornali - ha provocato 800 morti.

Onorevole Ministro, la ringrazio per la sensibilità istituzionale e per il tempo che dedicherà ad ascoltare il mio intervento, sperando non sia impegnato in conversazioni internazionali. La ringrazio per la sensibilità istituzionale che l'ha portata a riferire questa mattina in Parlamento, nonostante il *tour de force* che in questi giorni e probabilmente anche nei prossimi dovrà continuare Finalmente, dopo silenzi, smargiassate, divieti, tentennamenti, mistificazioni e bugie - colleghi, tante bugie - pensavamo questa mattina di capire su quale linea retta il Governo si stesse muovendo. però, questo è un Governo barcollante tra una vena sottile di xenofobo razzismo e azioni umanitarie spesso solo annunciate a parole, ma mai perseguite nei fatti.

Mi rendo conto che essere Ministro di centrodestra, in un Governo fortemente indebolito dai comportamenti di una maggioranza ossessivamente asservita ai bisogni del plurimputato Berlusconi, non deve essere facile.

ma umanamente mi è simpatico. Oggi però lei è venuto qui per dichiarare il fallimento completo delle politiche sull'immigrazione.

non convince, né sotto il profilo politico né sotto quello umanitario, né dal punto di vista della sicurezza e del rispetto delle garanzie costituzionali. È giusto che gli italiani sappiano la verità, Ministro, nonostante un'informazione, non solo quella del servizio pubblico, sempre più spesso teleguidata per non fare neppure filtrare la realtà dei fatti. Politicamente è stato squallido affidare il respingimento dei migranti ad un dittatore sanguinario come Gheddafi, che recuperava chi sfuggiva da fame, miseria, persecuzioni e guerra per portarlo in veri e propri campi di concentramento, dove

perché avete fatto fare un lavoro sporco alla stessa persona che oggi avete scaricato improvvisamente per cercare di riconquistare un minimo di credibilità internazionale; quella stessa persona che alcuni di voi, veramente in modo squallido**,** pretendevano venisse a parlare in questa sacra Aula del Senato. Non pensa, onorevole Ministro, che tutti i comportamenti del suo partito di appartenenza, forse per squallidi calcoli elettorali, abbiano arrecato danni incalcolabili all'Italia? È da mesi che ella afferma la possibilità di flussi biblici e che mai, con l'accordo Stato-Regioni-enti locali, avreste avuto problemi, come ha dichiarato anche il 3 marzo 2011, quando sfoggiava sicurezza e tranquillità. La verità invece è che è fin troppo evidente il pressapochismo con cui il Governo - sono veramente dispiaciuto nel constatare che soltanto la Lega Nord affronti a viso aperto un problema, perché gli altri sembra se la siano data a gambe

Ma è possibile che da dicembre ad oggi, nonostante la sua preveggenza, un Paese straordinario come l'Italia, potenza mondiale, non sia stato capace di trovare una una dignitosa sistemazione ai migranti? Chiamiamoli così, poi capiremo se sono profughi o clandestini, perché oggi non siamo ancora nelle condizioni di

Impreparazione o malafede? Come spiegare questo aumento di profughi, avvenuto senza un criterio di smistamento su Lampedusa? Signor Ministro, allora avete consentito che questo problema si esasperasse per poi smistare tutto smistare tutto e tutti sulle Regioni meridionali? E non mi dica che questo non è un calcolo - un po' cinico - della sua parte politica:

Purtroppo il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi: la situazione vi è sfuggita di mano, oggi provate a coinvolgere le Regioni e gli enti locali. Ho tra le mani questa mezza paginetta di intenti firmata

purché si capisca che in questo Paese nel 2010 vi sono state soltanto 10.000 domande di asilo politico, la Francia ne ha incassate 52.000, la Germania 49.000, la Svezia 32.000, la Gran Bretagna 24.000, il Belgio 26.000: non può entrare in crisi l'Italia per questo piccolo, grande flusso di migranti, che abbiamo il sacrosanto dovere di accogliere, con la sicurezza

dove andranno? È evidente, signor Ministro, lo sappiamo: per questo non ci convince quando sospende i diritti dei parlamentari. Se la collega Poli Bortone parla

immediatamente quella circolare e a farlo presto, altrimenti i parlamentari - e le parlo per me - entreranno clandestinamente all'interno delle

di sé. Signor Ministro, la stima *bipartisan* che la riguarda è un patrimonio che lei può certamente vantare e che le consiglio di spendere bene anche in futuro al servizio di questo Paese. Conosco anche la sua appartenenza politica e la rispetto ma, signor Ministro, se in questa vicenda lei fosse stato un po' meno uomo della Lega

Sono i prezzi che si pagano, in politica, nelle campagne elettorali: una dose di populismo, scelte che hanno segnato forse troppo. Oggi vi è meno bisogno, forti come siete, di caratterizzarvi su queste linee e schematismi ideologici, anche perché il tema dell'immigrazione è talmente grande che non può essere contenuto

politico. Cosa voglio dire con questo? Oggi lei ci ha detto in modo incerto fondamentalmente che avete cambiato strategia, che dalla linea dei respingimenti e dell'evocato blocco navale immaginato sulla base di un documento dell'Unione europea che non esisteva state ragionando in termini molto più flessibili, utilizzando l'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione in questa forma transitoria, ricorrendo a questa negoziazione con l'Europa tanto vituperata, che oggi diventa l'elemento di riferimento. Ma vorrei dirle, signor Ministro,

a quella vicenda che lei ha raccontato in modo quasi virtuoso: il caso di Mineo. Se Mineo sta cominciando a funzionare anche nel rapporto con il territorio, va dato atto anche a un onesto dirigente del Ministero dell'interno, il prefetto di Catania, che ha compiuto un'opera assolutamente apprezzabile di conciliazione degli interessi in campo, compresi quelli territoriali, chiedendovi anche di non mandare tunisini a Mineo come stava accadendo nella fase critica dell'emergenza. Stavate snaturando questo campo di Mineo che, come raccontano i radicali, è stato caricato svuotando tanti altri campi per farlo diventare il fulcro dell'accoglienza rispetto ai rifugiati politici. quando avete mandato i tunisini a Mineo da Lampedusa il campo è stato snaturato, con rischi anche di conflitti interni e con i problemi di sicurezza e di ordine pubblico all'esterno.

per adesso lo riconducete soltanto ai profughi che sono in numero molto limitato. Ma quel tema riguarda tutti i migranti che ad oggi gravano pesantemente ancora nelle Regioni meridionali, perché è evidente dal suo racconto che ancora oggi non avete individuato un solo sito, né in Lombardia, né in Veneto, né in Emilia, né in Piemonte. Ne avete individuato uno a Ventimiglia che si spiega molto bene, perché lì è l'ultimo passaggio per la Francia, e questo progetto sperimentale con la Toscana. Avete cambiato strategia, e ve ne diamo atto. Lo ha detto stamattina in toni morbidi, abbassando di molto il il tono della comunicazione. Questo è l'elemento che io colgo questa mattina anche delle agenzie: è il rapporto di collaborazione istituzionale, questa apertura alle Regioni, questo piano nazionale. Però il piano non esiste ancora, lei non ce lo ha comunicato, non ci ha detto come sarà definito

il timore di una ricaduta elettorale condiziona troppo il Governo, e lei in modo particolare. Per questo, signor Ministro, proprio per la stima *bipartisan* che

Concludo con Lampedusa. Non utilizziamo i territori deboli per le partite della politica, perché Lampedusa è stata utilizzata per sovraccaricare drammaticamente la situazione, e oggi l'isola deve essere risarcita, ma non con le chiacchiere del Presidente del Consiglio sulle ville che comprerà a Lampedusa, ma con i fatti:

Signor Ministro, sia il garante di questo Governo quantomeno nel rapporto con l'isola di Lampedusa, che ha pagato un prezzo tutto alla politica. *(LNP)*. Signor Presidente, cari colleghi dell'opposizione, a scanso di equivoci e per chiarezza, noi diciamo grazie al ministro Bossi per aver saputo efficacemente interpretare il pensiero di milioni di cittadini italiani. Grazie,

Diciamo grazie al ministro Maroni, a cui va la nostra massima solidarietà per il vile gesto di questa mattina alla Camera dei deputati, che qui nessuno ha ricordato. Grazie, ministro Maroni. Di fronte alle tragiche notizie che giungono dal confine più meridionale della penisola, acquista un particolare significato la presenza in quest'Aula del Ministro dell'interno, non solo per il ruolo che, che, istituzionalmente, è chiamato a svolgere in simili frangenti, ma anche in virtù dell'impegno profuso nella drammatica emergenza degli sbarchi clandestini sull'isola di Lampedusa e dei risultati ottenuti. Così, mentre esprimiamo il cordoglio del nostro Gruppo per le centinaia di vittime dell'ultima strage in mare, ci reca conforto apprendere che gli accordi raggiunti dal titolare del Viminale con il Governo della Tunisia porranno fine, come da auspicio, all'ecatombe che nel Canale di Sicilia è già costata 800 vite in appena tre mesi. Una strage immane, che ci induce a contrastare con ancora maggiore determinazione certe posizioni di irresponsabile istigazione all'immigrazione clandestina, dietro le quali si celano speculazioni politiche e finanziarie:

a mantenere basso il livello salariale, inflazionando l'offerta di braccia sul mercato del lavoro. E ancora, nell'attuale contingenza è echeggiata da più pulpiti la consumata esortazione all'accoglienza universale, principio di tale insensatezza che nella sua applicazione sostanziale dovrebbe condurci a spalancare le porte a un miliardo e mezzo di persone, perché tanti sono i poveri del mondo, e Siamo nel paradosso della demagogia, ma effettivamente, oltre a fulminare accuse di razzismo nei confronti di chi predilige il buonsenso al buonismo, la sinistra non è mai andata. *(Commenti dal

ai posti di lavoro e nell'aiutare a casa loro i popoli in via di sviluppo, due binari in grado di condurci fuori dalla cappa dell'immigrazione concepita come pericolo. E mi rammarico sinceramente che il sostegno alle popolazioni del Terzo mondo sinora non abbia conosciuto tutta la spinta indispensabile. D'altro canto, proprio la necessità di prevenzione e regolamentazione dei flussi migratori si è rivelata terreno idoneo a gettare le basi per un inedito modello di cooperazione: è avvenuto così nei rapporti con la Libia, sposando vantaggiosi accordi economici alle nostre esigenze di ordine e sicurezza; accade ora con la Tunisia. Anzi, da quest'ultima intesa emerge un aspetto di particolare interesse: la disponibilità del Governo tunisino al rimpatrio dei propri immigrati clandestini. Occorre riconoscere al ministro Maroni di aver realizzato una sorta di quadratura del cerchio, poiché non era semplice far accettare a un Paese ancora in fermento il recupero di un gran numero di soggetti insoddisfatti, dunque potenzialmente sovversivi o perlomeno inquieti. Tale considerazione spiega forse la richiesta del Governo di Tunisi di procrastinare nel tempo il rientro dei circa 25.000 suoi cittadini sbarcati a Lampedusa quest'anno, mentre si impegna a impedire nuove partenze. Importante, in tale contesto, il ruolo svolto dal Gruppo Lega Nord a Strasburgo, con la presentazione con la presentazione di una relazione approvata dal Parlamento europeo in cui si raccomanda ai Governi di assistere il nostro Paese e si sollecita l'attivazione del meccanismo di solidarietà previsto dai trattati, compresa la direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea degli sfollati. Si apprende, poi, dell'accordo Governo-enti locali finalizzato all'equa distribuzione su tutto il territorio nazionale del fardello migratorio: teniamo conto che il 90 per cento dell'immigrazione extracomunitaria è già al Nord, con i relativi costi economici e sociali. tutti elementi che inducono a considerare come la situazione di eccezionale gravità seguita ai rivolgimenti nel Nord Africa e all'insurrezione libica sia stata affrontata e gestita efficacemente. Concludo, signor Presidente, e, saltando qualche passaggio del mio sottolineare l'importanza che la temporaneità dei permessi non dia luogo a regolarizzazioni di sorta, affinché non si sancisca un meccanismo distorto di legittimazione dell'illegalità ed emulazione. In questi giorni, inoltre, abbiamo assistito sui media all'assimilazione dello *status* del profugo a quello del clandestino: crediamo occorra la massima chiarezza su queste figure, affinché dignità e diritti dei rifugiati non vengano usurpati da semplici profittatori, nei cui confronti deve scattare la prassi del respingimento. La demagogia, insomma, faccia un passo indietro, a tutto vantaggio dell'oggettività. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro dell'interno, ho pensato molto a che taglio dare a questo intervento, e mi permetto di dire che vorrei un po' disancorarmi dagli ultimi episodi d'Aula e dalle ultime forzature. Così come, lo dico al senatore Bodega, con assoluta chiarezza, come abbiamo fatto alla Camera, noi ci dissociamo assolutamente dal cartello che è stato esposto in quell'Aula. *(Applausi dai Gruppi* *PD, PdL è la disgrazia avvenuta al largo delle coste di Lampedusa, in nessun modo riconducibile a responsabilità del Governo italiano, che, anzi, che, anzi, è intervenuto con le motovedette e con altri mezzi per prestare soccorso. Chiedo soltanto ai colleghi della Lega di pensare al fatto che questo mare, che ci è sembrato nei primi mesi di quest'anno poter tornare, chissà, forse in torno di tempo non troppo lungo, un luogo come era secoli fa in cui le parole democrazia, pace, relazioni fra i popoli, erano improntate a regolarità e ordinarietà, in cui c'erano queste parole comuni, registra anche in una tragica metafora il massimo della negazione di quella speranza con gli ormai migliaia di morti che stanno facendo del Mediterraneo un'enorme fossa di corpi e di dolore. Le dicevo, signor Ministro, che ho esitato a lungo a scegliere la chiave perché - me lo lasci dire - il clamoroso fallimento delle politiche che sono state per quasi due mesi poste in essere, con ambiguità, contraddizioni, errori, mistificazioni, silenzi e omissioni dal Governo, avrebbe potuto oggi offrire una prateria. Ma noi siamo il più grande partito dell'opposizione e il secondo partito del Paese, e devo dire che oggi l'ho sentita imbarazzato, come non dovrebbe essere un Ministro dell'interno, molto attento a dire e non dire, a non irritare i colleghi della Lega, che infatti per primi hanno ringraziato il ministro Bossi per la sua famosa espressione che, essendo una signora, non ripeto. L'ho vista imbarazzato, e l'Italia tutto può essere in questo momento, tranne che essere presa da imbarazzo, se peraltro vuole far valere in tutte le sedi, a cominciare da quelle internazionali, il peso della propria autorevolezza e anche delle proprie pretese. Credo dunque che oggi dobbiamo venire a un giudizio assolutamente inclemente su quella che è stata la prima gestione di questa crisi. Oggi lei ha messo i fatti in ordine con molte omissioni e con qualche forzatura sulle quali tornerò, signor Ministro, e dalla lettura della sua relazione e ad ascoltare le sue parole pare che tutto sia andato liscio come l'olio, ma così non è stato. Le immagini di Lampedusa, ma non solo, le immagini di Manduria, che le televisioni hanno trasmesso in tutto il mondo, danno invece il segno di un fallimento, che è figlio di una tragica incapacità di scegliere politicamente che atteggiamento tenere: troppo forte è il ricatto della Lega. E mentre c'era la tentazione, che in qualche momento si è manifestata con evidenza, signor Ministro, di fare di Lampedusa una bomba, il caso, usando corpi anche di minori, spesso abbandonati, senza cibo, senza cure mediche, senza nessuno di quei presidi che servono per assicurare un'esistenza minimamente dignitosa; mentre non si capiva di che natura fossero questi centri in cui venivano stipate le persone; mentre troppo poche forze dell'ordine, con disposizioni del tutto contraddittorie, procedevano, non procedevano o procedevano male ai primi adempimenti dei centri di prima accoglienza (l'identificazione,

mentre tutto questo accadeva e non si capiva che cosa stesse succedendo; mentre qui il ministro Frattini vedeva che la maggioranza rifiutava di approvare le sue conclusioni perché, per esempio, egli aveva dato del Consiglio dei ministri europeo del 21 marzo una lettura propria, che era quella dell'utilizzo dei mezzi navali dei Paesi europei per opera di protezione umanitaria, e invece i colleghi della Lega volevano leggerlo e interpretarlo come possibilità di utilizzarli come blocco navale; mentre si susseguivano dichiarazioni in libertà sulla necessità di adoperare i vagoni per portare in Francia coloro i quali arrivavano in Italia o il filo spinato; mentre si irridevano coloro che sbarcavano considerandoli, come ha fatto il governatore del Veneto, quelli che arrivano con i jeans griffati; mentre tutto ciò accadeva, io capisco quale sia stato lo stato di confusione, e probabilmente di tensione e di conflitto, che si è registrato all'interno del Governo sulle scelte da fare, ma questo è stato il fallimento dell'Italia, oltre che della politica del Governo. Eppure, cosa fare era chiaro. Lei oggi ha ricordato più volte - e io credo che in questo modo abbia fatto opera di verità - altri interventi fatti in altre epoche da altri Ministri di altri Governi. Ha ricordato due volte il ministro dell'interno Giorgio Napolitano e la sua politica perseguita con grande attenzione

ed è stata interpretata male l'offerta di collaborazione che c'era in quella richiesta. Eppure gli strumenti ce li avevate tutti, però si devono affrontare senza ambiguità, signor Ministro: senza ambiguità. degli esempi, per comprenderci, cercando di tratteggiare quella che potrebbe essere una politica che, piano piano e con fatica, per necessità, state cominciando ad abbozzare. Vorrei dirvi, comunicandovi un'esperienza che conoscete, ma che fate finta di non conoscere, come potrebbe essere.

essere in possesso di un titolo come il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 20 non è sufficiente per entrare in altri Paesi europei. Diciamolo! E se c'è da fare qualcos'altro facciamolo, è importante farlo. Così come è importante dire che ovviamente non tutti i soggetti che restano sul territorio nazionale andranno andranno via, ma resteranno qui. Quindi bisognerà, con l'accordo delle Regioni, fronteggiare questa situazione. dell'accordo con le Regioni noi la trasporremo in una mozione che sottoporremo anche al voto dei colleghi della Lega, perché vogliamo che sia chiaro qual è la politica dell'Italia su tale questione.

perché così non può non essere, che questa politica dei rimpatri deve essere rispettosa della direttiva 2008/115/CE, che voi non avete voluto recepire, che è entrata in vigore necessariamente il 24 dicembre, che oggi prevale sulla legge nazionale e rispetto alla quale lei il 17 ha predisposto una circolare che non la rispecchia fino in fondo. È una direttiva europea sulla base della quale tutte le procure della Repubblica d'Italia

Questo, a dimostrare che andare dietro alle ambiguità e alle reticenze sulle politiche europee è un errore tragico.

della direttiva del 2008. È un fiato corto, quello che vi ha spinto in questi mesi di governo. Poi, certo, bisognerà fare prevenzione: siamo assolutamente d'accordo. Gli accordi con gli altri Paesi? Siamo assolutamente d'accordo. Questa politica l'abbiamo inaugurata noi con il Governo Prodi e l'Albania: siamo d'accordo. Si deve fare la cooperazione internazionale? Ma allora ci vogliono le risorse, e non bisogna respingere tutti gli emendamenti che vengono dal Parlamento

alla gola, e non anche quando dall'Europa potrebbe avere, con rispetto delle decisioni, un riconoscimento che aiuti a dare forza al nostro Paese e a dire, in un momento come questo, che l'Italia non si è mai sottratta,

di meno - ci sia uno strumento utile serio. E quando si dice «su tutto il territorio nazionale», colleghi della Lega, si dice «su tutto il territorio nazionale», perché la solidarietà su questo punto non la si può pretendere per l'Italia e non pretenderla per tutte dal Gruppo PD)* e per tutti i cittadini, di qualunque comunità, che si trovino nelle condizioni di prestare accoglienza! Bene, questo accordo è un passo. Noi siamo un partito serio, ci assumiamo sempre le nostre responsabilità quando siamo al governo: oggi con i nostri amministratori e con i nostri presidenti di Regione siamo in grado di corrispondere alla responsabilità che ci viene richiesta. Ma dall'altra parte pretendiamo che sia assicurata la stessa identica responsabilità: non soltanto da lei, ministro Maroni, che molto spesso

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, in primo luogo anche il Gruppo del Popolo della Libertà esprime in questa Aula il proprio cordoglio per la tragedia che si è verificata nei giorni passati nel Mediterraneo. proprio nel Mediterraneo, l'Italia in tutti questi anni abbia fatto fronte a numerose emergenze umanitarie e vogliamo auspicare, come Gruppo, che Malta possa avere una politica di maggiore collaborazione, di maggiore attenzione e sollecitudine, perché anche nel passato - Malta, che pure ha una competenza molto ampia nell'area mediterranea, spesso forse non adeguata ai mezzi navali e alle possibilità di controllo, possa rendersi conto di queste emergenze e condividere, appunto in quel consesso europeo tante volte questa mattina richiamato, interventi umanitari e capacità di affrontare emergenze. La situazione che stiamo affrontando in questi giorni deriva da vicende di natura storica: la storia si è rimessa in cammino nel Mediterraneo. Se non partiamo da questa premessa, facciamo considerazioni assolutamente fuori luogo, come quelle che anche poc'anzi ho ascoltato da alcuni banchi. banchi. Nel ringraziare il Governo, il ministro Maroni e il presidente Berlusconi per gli interventi che in questi giorni hanno promosso anche in Tunisia, nel dialogo con le nuove autorità, voglio rivendicare la validità della politica attuata in questi anni da questo Governo nell'area mediterranea in condizioni ordinarie. Cari colleghi, quando governavano alcuni che adesso fanno la voce grossa, gli sbarchi erano arrivati ordinariamente a livelli inauditi, in condizioni disumane che nessuno voleva poi seguire con l'attenzione e con la commozione che talvolta si ostenta ora. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Era un'emergenza quotidiana, il centro di Lampedusa era diventato un luogo dove ogni giorno si verificavano situazioni complesse, difficili, oltre i livelli accettabili. La politica realizzata dal Governo Berlusconi, con l'impegno del ministro Maroni e dell'intero Esecutivo, ha portato ad un maggior rispetto dell'Italia, ad un dialogo con altri Paesi e con i Governi che c'erano,

tre mesi fa, che Mubarak avrebbe lasciato la guida dell'Egitto, che Ben Ali, con le proteste popolari, avrebbe lasciato la guida della Tunisia, che in Libia scoppiasse un conflitto, una situazione che sta impegnando anche l'Italia. Ne abbiamo già discusso e ho già ricordato in quest'Aula come ho trovato tanti tardivi laudatori della

La storia si è rimessa in cammino e non c'è dubbio allora che dobbiamo affrontare questa emergenza in maniera adeguata, distinguendo profughi da clandestini.

altrove arriveranno quei profughi che già nei giorni scorsi l'intesa con le Regioni ha determinato debbano essere accolti da tutti. Il problema qual è? Che molti altri non sono profughi che fuggono da situazioni di guerra; sono persone che approfittano della storia che si è rimessa in cammino e della rivoluzione che ha travolto governi e assetti

scappano da un conflitto, non è facile accertarlo. E allora, di fronte alle emergenze della storia, ci si attrezza: con l'accoglienza umanitaria per i profughi, affrontando con realismo le situazioni che si sono verificate anche dalla Tunisia e riprendendo le fila del dialogo con i Governi che si stanno faticosamente costituendo. Il ministro Maroni - non credo di rivelare un segreto di Stato - mi ha detto giorni fa che le autorità che ha incontrato già gli hanno annunciato che pochi giorni dopo sarebbero state sostituite da altre; e le autorità che stanno governando la Tunisia - era scritto anche sui giornali - hanno già annunciato che alle elezioni non si candideranno. Quindi, già sappiamo che durante l'estate, quando si voterà in Tunisia, gli interlocutori saranno altri ancora. Tutto questo crea problemi e difficoltà per i riaccompagnamenti e per il rispetto delle regole. Ma il nostro obiettivo è e resta che i clandestini tornino a casa loro, perché non possono entrare illegalmente nel nostro Paese.

faticose trattative durate ore e ore, con interlocutori che su un dettaglio o su una parola cercano di imbastire un lungo confronto. Dovremo affrontare spese, dotare di mezzi di controllo che forse già nel passato concedemmo, ma che devono essere rinnovati. Ebbene, in questo contesto, se la storia si rimette in cammino, l'Europa non può stare ferma. Più grandi sono le emergenze, più grandi devono essere le convergenze. Peraltro - lo dico per inciso - fa bene il Governo ad applicare l'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione e ad invocare la direttiva 2001/55/CE, su cui c'è un contenzioso: le persone che disporranno di questo permesso temporaneo potranno muoversi nell'area Schengen? A nostro avviso sì, e non è un'opinione politica, bensì un'opinione giuridica che il Ministero dell'interno, anche oggi nel confronto con il Parlamento, attraverso le parole del ministro Maroni ha ribadito e motivato. Poi è chiaro che la Francia non è entusiasta e quindi controbatterà questa tesi con suoi argomenti e suoi cavilli. Ma vi è anche da dire che la via del dialogo, del confronto e del rispetto dell'Italia si è dimostrata con la richiesta venuta dalla Francia, dal presidente Sarkozy, di un vertice bilaterale che avverrà nei giorni prossimi. Poi sono tutti umanitari per conto terzi,

l'Italia deve essere sostenuta, che il programma Frontex deve essere intensificato, che l'operazione congiunta Hermes 2011 è stata lanciata dopo che l'Italia ha chiesto aiuto alla Commissione europea. In altri termini, si riconosce da parte della Commissione europea e del commissario Malmström quello che è un dato geografico: siamo il primo approdo del Mediterraneo. La nostra posizione geografica e la nostra posizione geopolitica ci rendono esposti ai rischi, ma ci danno anche delle opportunità. Ecco perché questo Governo ha sviluppato una politica nel Mediterraneo che ha portato maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici dell'Italia, che dipendono dall'estero, e ha portato ad un azzeramento degli sbarchi e dei flussi di clandestini. Ed io mi auguro che la nuova stagione di libertà, di democrazia, che dovrebbe percorrere l'area mediterranea ci consenta di avere Governi che assicurino il rispetto di quelle intese, il blocco delle partenze, la lotta ai trafficanti di morte. nell'esprimere il cordoglio nei confronti delle vittime di questa grande tragedia della storia dobbiamo rinnovare la denuncia per quegli omessi controlli che consentono ai trafficanti di persone di realizzare il loro turpe commercio ed esporre al rischio di morte centinaia e centinaia di persone. Questo non va mai dimenticato, per cui quei Governi che nasceranno e stanno nascendo nascendo devono avere il rispetto e la collaborazione dell'Italia e della comunità internazionale, ma devono anche imporre legge ed ordine all'interno dei loro confini.

e delle richiamate direttive europee; una politica di accoglienza per i profughi, ma anche una politica di fermezza nei confronti dei clandestini. L'Italia farà sentire la sua voce in Europa, con i nostri confinanti europei, ma anche nei confronti della Tunisia e di altre Nazioni. Abbiamo realizzato in condizioni normali la migliore politica di sicurezza e di contenimento dell'immigrazione degli ultimi anni. Dobbiamo affrontare una emergenza storica: il senso di responsabilità dovrebbe vedere tutti sostenere la giusta e corretta azione del Governo nel Mediterraneo

seria e, di fronte anche all'emergenza della storia, un Governo capace ed energico saprà riaffermarla.

con un atto di impiccagione, ma anche con un atto di strangolamento compiuto da altri. Per tutti questi motivi, sarebbe veramente necessario che il Governo risponda rapidamente a questa interrogazione che - lo ricordo - è soltanto l'ennesima, quanto la situazione delle carceri italiane richiederebbe un'attenzione maggiore di quella che fino ad ora ha prestato il Governo. Sicuramente il fatto è in sé grave, e mi pare che né la seconda né la terza carica dello Stato abbiano avuto modo di partecipare ad una decisione così pesante, né tanto meno di stigmatizzarla. Non si può neanche avere il testo della circolare in questione.

È possibile negare a un parlamentare l'accesso a un luogo pubblico o di interesse pubblico come sono questi luoghi? se si ritiene che siamo ancora una volta al di fuori della legge a seguito di misure emergenziali, almeno che si sappia il perché

Grazie

Grazie